ottenere, anche per i nostri cittadini, quelli che ascoltano e che hanno condotto una battaglia insieme a noi a Fondi, la soluzione di questo problema. Non è stato ancora sciolto il Comune di Fondi: approfondirò quando ve ne sarà

Si tratta del caso del trentino Enrico Forti, detenuto negli Stati Uniti da dieci anni, a Miami, condannato all'ergastolo per un omicidio che giura di non aver commesso. D'accordo con la famiglia, questa mattina

ogni ricorso per via ordinaria è stato respinto: solo la Corte federale ora può decidere di riaprire il processo e pare che solo il presidente Obama possa riuscirci. Segnalo questo ai molti colleghi che firmarono un'interrogazione in materia: se vogliono far pervenire un segno di pressione verso il Presidente del Consiglio, questo è il momento. Stamani invierò a tutti copia della lettera inviata al presidente Berlusconi. *(Applausi del

ha dichiarato, in seguito alla propria elezione a parlamentare europeo, di voler rassegnare le dimissioni da senatore della Repubblica, con decorrenza dalla prima seduta del Parlamento europeo, che avrà luogo il 14 luglio 2009. Trattandosi di dimissioni originate da motivi di incompatibilità e conseguenti ad un'opzione, l'Assemblea non può che prenderne atto. Pertanto le dimissioni dispiegheranno effetto dal 14 luglio 2009. Credo di interpretare

Signor Presidente, il senatore Berselli ed io ci rimettiamo alla relazione scritta per una compiuta analisi del provvedimento che dà attuazione alle intese internazionali raggiunte in materia di lotta alla pirateria. In particolare, il provvedimento disciplina l'esercizio della giurisdizione penale da parte dall'autorità italiana per gli atti di pirateria posti in essere al largo delle coste somale, dove è operativa la missione militare europea Atalanta cui l'Italia partecipa attivamente. Questo provvedimento, che è stato approvato con voto unanime dall'altro ramo del Parlamento, è stato esaminato dalle Commissioni riunite giustizia ed esteri, registrando anche qui in Senato il consenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari. Raccomandiamo quindi una sollecita definizione dell'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto che è un tassello significativo dell'azione che vede l'Italia impegnata sui più delicati scenari internazionali insieme agli altri Paesi dell'Unione europea.

Dichiaro aperta la discussione generale.

con la formula prendere o lasciare, tutto ciò che magari avremmo sostenuto ma che allo stesso tempo avremmo voluto approfondire. Quest'anno tutto ciò non avverrà e non sarà possibile avere un dibattito sulle missioni italiane all'estero ma, per l'appunto, è stata sfilata dal pacchetto la nostra partecipazione alla missione

però, si limita, se non altro nel dettato di quel documento, la presenza di una forza internazionale a scorta, difesa e protezione delle imbarcazioni del Programma alimentare mondiale: quindi qualcosa di leggermente diverso in riferimento alla lotta alla pirateria.

commerciale del trasporto di qualsiasi tipo di beni, ma in particolare dei due terzi del petrolio prodotto in Medio Oriente, sia nella penisola arabica

Un giornale che credo non si sia mai risparmiato nella promozione della mano ferma, il "The Wall Street Journal", quando l'anno scorso si era al picco di attacchi contro imbarcazioni che trasportavano sia petrolio che - caso clamoroso - addirittura una trentina di carri armati sovietici destinati al Kenya, dove

restituito a seguito del pagamento di riscatti o di iniziative di diplomazia muscolosa che non necessariamente hanno implicato l'utilizzo di danari,

fregate e comunque dispiegando la propria forza di terra, di cielo e di mare (credo che si debba proprio dire, perché non si tratta soltanto di navi) in quella parte del mondo. In nessuno dei passaggi relativi a questo esercizio ci si è posti il problema da parte europea di cogliere l'occasione, come ho cercato di dire ieri in relazione al dibattito sul modello nazionale di difesa, di organizzare una presenza sotto la bandiera dell'Unione europea, cioè di coordinare un comando sul Corno d'Africa, magari in forma di esperimento, visto e considerato che il numero di di cargo che corrono questo rischio è probabilmente maggiore all'1 per cento ma si sa che, proprio perché si tratta di pirati molto selvaggi, per non dire selvatici, soltanto l'1-2 per cento viene interessato dai loro attacchi; ripeto, si sarebbe potuto tentare di coordinarsi sotto la bandiera con le 12 stelle e invece si è deciso di non farlo. accelerato un processo di inclusione, all'interno di questo tipo di iniziative, della Marina russa e anche della Marina cinese, con una sorta di

è lecito utilizzare qualsiasi tipo di mezzo per debellare la pirateria, ma allo stesso tempo sappiamo che, negli ultimi quarant'anni, sono stati adottati strumenti di

L'altra questione che non si è voluto prendere in considerazione, posto che nessuno mette in dubbio la buona fede di questo esercizio, è che ci si va ad interessare di un Paese, la Somalia,

vantare il controllo di tutto il territorio riconosciuto secondo il diritto internazionale come Somalia. Questo non è stato fatto per tutta una serie di motivi. Innanzitutto, negli anni scorsi, grazie all'insistenza dell'amministrazione Bush, si è ritenuto che il Corno d'Africa fosse una delle

ad una parte del Ruanda che confina con il Congo e che continua ad essere armata malgrado la presenza delle Nazioni Unite e l'attività dei vari tribunali e corti penali internazionali o internazionalizzate che da anni esercitano la propria giurisdizione in quegli ambiti. è quindi cercata la soluzione militare rispetto a quella che avrebbe potuto iniziare ad essere una soluzione politica. Sappiamo che quando si discute la conversione di un decreto-legge

che riprende ciò che avevo tentato di sollecitare l'anno scorso quando, per la prima volta, fu inclusa la partecipazione italiana alle missioni internazionali

che, contrariamente al resto del Paese, è riuscito a mantenere un minimo di presenza e di lavoro di istituzioni nazionali nazionali ed un minimo di presenza e di godimento di diritti civili e politici, con tutte le problematicità che può avere un Paese non soltanto circondato dal nulla dal punto di vista politico-istituzionale ma anche fortemente povero. Tale zona, quindi, contrariamente a quanto ho cercato di affermare in precedenza, e cioè che a questo tipo di problemi bisognerebbe rispondere politicamente ancor prima che militarmente, avrebbe potuto essere utilizzata come base di partenza per alcune navi della flotta internazionale. di prendere in considerazione sia la possibilità di sondare i *partner* europei più attivi nella lotta alla pirateria, come Germania e Francia, che hanno già stabilito dei contatti con le autorità - definiamole anche in senso, a considerare forme di collaborazione con il Somaliland nel contrasto efficace alla pirateria e nella ricerca della stabilizzazione della Somalia non escludendo attenzione all'esercizio democratico praticato in quella zona. che nel mese di novembre il Somaliland eleggerà un presidente ed io credo che, magari inviando una delegazione informale di parlamentari, si possano unire i due aspetti della lotta alla pirateria da una parte e del recupero della stabilizzazione di un Paese come la Somalia dall'altra, attraverso la promozione di quel minimo di democrazia e di Stato di diritto che i somalilandesi sono riusciti a mantenere negli anni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di riassumere il mio intervento e chiedo di depositare il testo integrale. La pirateria navale - quale attività illecita posta in essere da organizzazioni criminali al fine

ossia di quella categoria di delitti particolarmente efferati nei confronti dei quali ogni Stato può, in linea di principio, esercitare la propria potestà coercitiva e punitiva, anche oltre i limiti ad esso normalmente assegnati dal diritto internazionale. Tali reati possono, per l'appunto, essere perseguiti e puniti da ogni Stato, anche in mancanza di un loro collegamento diretto o indiretto con la comunità territoriale ad esso sottoposta. Inoltre, in relazione a questi reati, è anche lecita la cattura dei rispettivi autori in alto mare, a norma del diritto consuetudinario. Negli ultimi anni tale efferato crimine, dalle radici dunque memorabili, è drammaticamente tornato alla ribalta funestando numerose spedizioni marittime e affliggendo, in particolare, specifiche nonché oramai tristemente note aree. Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2008 si sono verificati nel mondo oltre 1.850 atti di pirateria, cioè quasi uno al giorno; da una decisa diminuzione di questi avvenimenti dal 2003 al 2006 si è assistito, nel 2007, ad un nuovo aumento della pirateria marittima su scala mondiale, *trend* che nel 2008 è cresciuto ulteriormente. In tale anno, infatti, la pirateria marittima ha raggiunto livelli senza precedenti,

Nell'ordinamento italiano il reato di pirateria navale è disciplinato dal codice della navigazione, più in particolare dagli articoli 1135 e seguenti, che punisce con la reclusione che punisce con la reclusione da 10 a 20 anni il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera che commetta atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero che a scopo di depredazione commetta violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera. Nello scacchiere somalo c'è un ruolo diretto dell'Italia: la forza navale NATO è schierata nelle acque territoriali del Paese africano per prevenire i sequestri di navi cargo che, tra gli altri, ha visto al comando il contrammiraglio Giovanni Gumiero. Le unità hanno un mandato in bianco dalle Nazioni Unite per impedire «con ogni mezzo» l'azione dei pirati, tanto da guadagnarsi lo scorso 16 dicembre la prima pagina del «New York Times». È sempre grazie all'intervento della marina militare italiana che lo scorso aprile è stato evitato il peggio ad una nave porta-container italiana, la Neverland, diretta in India e attaccata nelle acque del Golfo di Aden di fronte alle coste somale da un gruppo di pirati armati di mitra e missili anticarro che le si sono avvicinati a bordo cinque barchini per darle l'arrembaggio.

appare tuttavia doveroso rilevare quanto autorevolmente avvertito durante il convegno del 28 novembre 2008 tenutosi a Genova sull'argomento «La pirateria: una guerra sul mare continuata con altri mezzi», nel corso del quale è stato evidenziato come il fenomeno è lungi dal potere «essere debellato con il solo contrasto in mare. La soluzione del problema risiede nell'eliminazione dei problemi alla base del fenomeno e, per quanto riguarda la Somalia in particolare, è da ritenere che - in assenza di una stabilizzazione delle istituzioni di governo di quel Paese (purtroppo ancora in preda all'anarchia ed alla guerra civile) - il mancato controllo del territorio consentirà il perdurare del fenomeno in tempi non brevi». **Testo integrale della dichiarazione per le azioni che sta svolgendo in questa zona, non solo sul piano più strettamente militare o navale, come abbiamo sentito e come con questo disegno di legge cerchiamo di incentivare al fine di inquadrare meglio la questione nello scacchiere internazionale e nella legislazione internazionale e nazionale,

*(PD)*. Signor Presidente, il provvedimento che discutiamo e che

in qualche misura desta stupore perché ci richiama a un vocabolario che sembrava far parte più dei nostri ricordi di infanzia e delle nostre letture giovanili che della situazione politica internazionale da affrontare nel nostro si tratta, come sappiamo, di un provvedimento importante, che affronta un fenomeno che si è via via sviluppato

il Golfo di Aden, passano gran parte delle merci, in particolare i prodotti petroliferi che transitano verso l'Europa e anche verso il nostro Paese. Com'è noto, da tempo la comunità internazionale si è organizzata per fronteggiare questo fenomeno. La missione Atalanta ha svolto e ha svolto e svolge in modo efficace la sua azione e il suo mandato; i primi risultati che oggi siamo in grado di valutare ci indicano il suo ruolo positivo. Naturalmente sappiamo anche che, stanti le condizioni attuali, non si tratterà di un fenomeno di breve periodo, destinato ad essere risolto esclusivamente sul piano del contrasto militare e attraverso quel tipo di intervento che la missione Atalanta Quello che la discussione di questa mattina mette in rilievo e ciò che in qualche misura sta dietro e sottende la nostra discussione è invece la difficoltà

la situazione internazionale. Quello che è successo in questi anni nelle regioni del Corno d'Africa e l'incapacità della comunità internazionale di offrire una soluzione nonostante i vari tentativi che sono stati effettuati, è forse la causa più importante che oggi

su questo provvedimento - una valutazione positiva - con la presentazione di un ordine del giorno che, oltre a chiedere al Governo di agire per rendere più trasparenti e più chiari i sistemi di trattativa, di concertazione e di definizione delle controversie irrisolte, pone un problema che riguarda in particolare il rapporto il Kenya, che ha un ruolo importante e con il quale è stato sottoscritto un impegno perché riceva le persone che vengono arrestate nel corso delle operazioni di pirateria. Nel corso di questa trattativa sono state date ampie garanzie sul trattamento delle persone arrestate. Non possiamo tuttavia dimenticare che il Kenya è uno dei Paesi nei quali la pena di morte, anche se da molto tempo non vengono praticate esecuzioni capitali.

questo problema e legittimando nuove preoccupazioni per il comportamento di questo Paese su tale materia, che, come sapete, è per noi tanto delicata e tanto importante ed è stata tanto oggetto di impegno dei diversi Governi italiani nei diversi periodi. Per questo, l'ordine del giorno G1 chiede che l'approvazione del provvedimento sia accompagnata da un impegno del Governo perché questi punti siano attentamente monitorati e si garantisca che in tutte le operazioni che riguardano il trattenimento, l'arresto e la detenzione di persone che il provvedimento che oggi approviamo comporta, siano rispettati quei principi costituzionali e quei riferimenti ai diritti umani che costituiscono un aspetto essenziale per

unanime. È doveroso ricordare ed evidenziare la rilevanza di tale fenomeno. L'annoso problema della pirateria ha origini antiche. Basti pensare che già nel 229 avanti Cristo i romani attribuirono al fenomeno una cornice giuridica *ad hoc* e fornirono a chiunque la legittimazione a combattere e, se possibile, a sterminare i pirati di allora. Oggi il problema si fa tanto più minaccioso quanto più strategico è il rapporto che lega i trasporti marittimi alle esigenze dell'economia

Già la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982, ratificata dall'Italia nel 1994, dichiarò la pirateria un crimine di carattere internazionale. In alcuni Paesi - e la Somalia sicuramente primeggia su tutti - il fenomeno negli ultimi anni si è aggravato. Nel 2008, come ha ricordato il collega della Lega Nord senatore Vaccari, vi è stato un incremento del 200 il numero stimato di questi predatori è passato da circa un centinaio ad oltre 1.600. Con il passare del tempo si consolida il concetto "pirateria uguale minaccia alla pace mondiale". in seguito all'*escalation* dello scorso anno, l'ONU ha emanato ulteriori risoluzioni, più forti e più decise, più decise, che autorizzano a perseguire e a contrastare con ogni mezzo i pirati, sia in acque internazionali che in acque territoriali, e che consentono l'aiuto e la scorta a qualsiasi unità navale, battente qualsiasi bandiera, quando questo aiuto venga richiesto. Va detto che il nostro Paese è stato il primo a prendere contromisure a ridosso del territorio somalo e merita ricordare l'efficacia della missione Atalanta. In futuro però l'azione, per poter produrre maggiori effetti, dovrà essere più incisiva, prevedendo, oltre alla fase della repressione, anche quella della prevenzione. distruzione delle basi logistiche a terra e l'isolamento dei pirati dalla realtà e dalla comunità di appartenenza; rendere sempre più difficoltoso il riciclaggio del bottino;

Un *report* delle Nazioni Unite del 2006 evidenzia che la Somalia, senza la presenza efficiente di una guardia costiera, sta diventando un mercato libero per tutti i pescherecci d'altura battenti bandiere di molti Paesi, quali ad quali ad esempio Spagna, Giappone, Corea del Sud. Tali pescherecci hanno operato lungo le coste somale in totale situazione di illegalità e senza alcuna licenza. La stima del saccheggio a danno della Somalia è di 300 milioni di dollari in pesca all'anno. Questo, evidentemente, accresce una situazione di povertà che rischia di sfociare proprio nel fenomeno della pirateria. La Somalia oggi è un Paese dominato dalle armi, dove non esistono regole e controlli, e questo vale soprattutto per il mare. Ecco perché l'opera di prevenzione appare oggi necessaria ed urgente. ed urgente. A fronte di quanto esposto si può già, in sede di discussione generale, anticipare un convinto consenso a questo provvedimento da parte Lega della Nord, anche in considerazione del fatto

Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve trattandosi di un provvedimento condiviso, anche se da tutti viene raccomandata una certa cautela, soprattutto sotto il profilo

L'intervento di un componente della Commissione giustizia si giustifica perché sostanzialmente la pirateria si configura come un crimine internazionale che rientra tra i cosiddetti *Treaty crimes*, vale a dire tra i comportamenti che la comunità internazionale percepisce come reati, classificati alla stregua di crimini proprio attraverso trattati.

tanto che - come è stato ricordato anche da altri colleghi - la pirateria costituisce uno dei più antichi illeciti, classificato tra le ipotesi dei cosiddetti *crimina iuris gentium*. La pirateria è disciplinata e dettagliata dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982, firmata a Montego Bay, agli articoli 100 e seguenti, che, con qualche modificazione, riproducono gli articoli 14 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 1958.

sia di fronte alle nuove minacce di penetrazione di integralismo islamico, sia di fronte a una minaccia di instabilità per il continente africano in generale. Non c'è dubbio che il nostro Paese deve avere un ruolo importante,

recinta la giurisdizione italiana per quanto riguarda la pirateria in danno di beni e uomini, limitandola ai soli casi in cui i fatti siano commessi a danno dello Stato, di cittadini o di beni italiani in alto mare o in acque territoriali, anche terze, e accertati nell'area in cui si svolge la missione Atalanta. Questo avviene attraverso la modifica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008. Peraltro, la preoccupazione riguarda il trasferimento di persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in base alle suddette azioni,

che il Governo vigili affinché il nostro partner, il Kenya, il Paese che si occuperà del giudizio e della detenzione di coloro che dovessero rendersi responsabili di atti di pirateria,

fondamentali, universalmente riconosciuti non solo sulla base dei trattati ma sulla base del diritto internazionale codificato al di là di norme scritte, che debbono assicurare la piena difesa e l'umanità dei trattamenti, evitando la tortura e la pena di morte per i detenuti. Con questa precauzione naturalmente il mio intervento è a favore del provvedimento

Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1 il relatore esprime parere favorevole, trattandosi del medesimo ordine del giorno presentato il 1° luglio scorso alla Camera dei deputati dall'onorevole Paolo Corsini

in quanto implica un riconoscimento implicito del Somaliland. Tutti conosciamo le vicende che hanno caratterizzato quella regione, però è altrettanto vero che dobbiamo non disintegrare l'unità territoriale e nazionale di quell'area, ma sostenere

in sede di discussione del disegno di legge n. 1652, considerata la partecipazione italiana alla Missione Atalanta,

a considerare forme di collaborazione con il Somaliland - in stretto raccordo con le istituzioni federali transitorie a Mogadiscio nel contrasto efficace alla pirateria e nella ricerca della stabilizzazione della Somalia non escludendo attenzione al buon andamento delle prossime consultazioni elettorali in quella regione. il relatore esprime parere favorevole,

In questi giorni il dibattito sul G8 ha nuovamente evidenziato un aspetto problematico che da sempre caratterizza l'Unione europea: la mancanza di una voce unica Tale deficit è ritenuto causa principale del mancato raggiungimento di risultati concreti nelle crisi internazionali, dalla Georgia all'Iran, per citare l'ultima, dove Francia, Germania e Italia hanno mantenuto posizioni distinte e anche per questo sono riuscite ad incidere poco o niente. In Iran continua la repressione, in Georgia le truppe russe non sono mai tornate sui confini di prima dell'invasione di Abkhazia e Ossezia. Per queste ragioni, a livello di dibattito politico sul G8, è fortemente appoggiata la creazione di una forza militare comune, nonché l'istituzione di un vero e proprio Ministro degli esteri europeo al posto della figura ambigua dell'Alto rappresentante per la politica estera, Javier Solana, il quale non a caso ha praticamente rassegnato le dimissioni, sconfortato dalla mancanza di mezzi e di incisività europea in politica estera. Cari colleghi, ecco perché accordi come quello che stiamo ratificando oggi, che vedono la partecipazione integrata delle forze europee, nell'ambito dell'azione comune 2008/851/PESC, volta alla repressione degli atti di pirateria al largo della Somalia, non possono che trovare l'Italia dei Valori favorevole. Questi sono i piccoli passi con i quali si procede verso una sostanziale unificazione della politica estera europea e delle sue Forze niente da eccepire, se non che la modifica che è stata fatta all'articolo 4 del decreto di rifinanziamento delle missioni internazionali, che limita la giurisdizione italiana ai soli casi in cui gli atti di pirateria vengano commessi a danno del nostro Stato, dimostra come prevalga una logica di autoreferenzialità che riduce in parte il nostro campo di azione, circoscrivendolo a fatti che riguardano soltanto il nostro "orticello".

il suo intervento. È anche umiliante per i singoli senatori, di sicuro per me, fare l'appello di quelli che non consentono di lavorare. Però, se è l'unico modo, si procederà

il mare ha sempre assunto un ruolo fondamentale nelle relazioni economiche, politiche e sociali tra gli Stati perché rappresenta la principale via commerciale. Le rotte marittime sono certamente un elemento di forza dei sistemi economici moderni, ma anche un elemento di vulnerabilità perché costituiscono il contesto ideale per il fenomeno della pirateria marittima. La lotta alla pirateria marittima a largo delle coste della Somalia e nell'Oceano Indiano ha assunto negli ultimi anni un ruolo importante nell'ambito delle politiche sulla sicurezza della navigazione marittima

In particolar modo, l'Unione europea ha attivato la missione Atalanta, decisa dal Consiglio europeo nel settembre 2008. Il Senato il 18 dicembre 2008 ha approvato un ordine del giorno unitario in cui si impegnava il Governo a cooperare a tutte le iniziative antipirateria e ad adottare sollecitamente provvedimenti diretti a consentire all'Italia di prendere parte alla missione navale dell'Unione europea nel mare prospiciente la Somalia. Uno dei problemi da risolvere nelle missioni antipirateria è la sorte dei pirati catturati, della nave e del carico. Si pongono spesso questioni delicate di concorso di giurisdizioni qualora, per esempio, la cattura avvenga nelle acque territoriali somale. L'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, che abbiamo convertito nella legge 24 febbraio 2009, n. 12, contiene le prime disposizioni *ad hoc* sulla pirateria marittima. Con il disegno di legge al nostro esame, di conversione del decreto-legge n. 61 del 15 giugno 2009, modifichiamo queste disposizioni per rendere ancora più efficace la lotta alla pirateria e dare attuazione all'accordo con il Governo del Kenya sul trasferimento in quel Paese delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria a largo della Somalia.

Al di là dell'esigenza di chiarire alcuni profili legati alla giurisdizione e di rispettare gli accordi internazionali sulla materia, è chiaro che questo provvedimento ha solo una portata di natura tecnico-giuridica e non ha altro tipo di presunzione. Quindi, l'unica considerazione che possiamo fare, oltre alla valutazione positiva del merito del provvedimento, è che comunque restano aperti tutta la questione relativa alla Somalia e il tema della garanzia e del rispetto dei diritti civili anche in Kenya, Paese chiamato a gestire i pirati che vengono

non soltanto perché si tratta sostanzialmente e in diritto di un atto dovuto, facendo seguito alle indicazioni del Consiglio dell'Unione europea ed anche del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; voterà a favore anche perché convinto della bontà del contenuto e della necessità di regolamentare una situazione giuridica interna che in questo momento è ancora monca. Si tratta, in effetti, di un adeguamento delle norme interne, sostanziali e processuali, ad una situazione storica molto delicata come quella che si sta osservando in uno degli scenari più a rischio dello scacchiere internazionale. In particolare, nel disegno di legge al nostro esame vengono precisati la fattispecie penale del delitto contestabile, quello di pirateria, ed i compiti delle forze di intervento ai fini della repressione penale. Il Partito Democratico, pertanto, conferma l'importanza e la necessità di adeguarsi alle norme del diritto internazionale sulla base del disposto della nostra Carta costituzionale

in merito alla tutela dei diritti fondamentali di ogni singola persona, per fare in modo che venga garantito che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante, compresa la possibilità per le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali di visitare, su loro richiesta, le persone trasferite. In questa ottica il Partito Democratico conferma il proprio voto favorevole.

ha indotto quello del Popolo della Libertà a concentrare nella dichiarazione di voto l'esposizione delle ragioni per cui con convinzione lo voterà. La pirateria, quella marittima in modo particolare, nella sua moderna accezione, al di là delle suggestioni romantiche che una certa narrativa per adolescenti può evocare in molti di noi, è un fatto di assoluta brutalità: rappresenta un evidente regresso culturale e al tempo stesso un pericoloso attentato alla sicurezza marittima nel trasposto di persone e cose.

la sua operatività all'estero. Quindi si è opportunamente provveduto ad un adeguamento delle norme interne ai fini di una migliore individuazione della giurisdizione nell'ambito della missione Atalanta, per quanto riguarda la competenza del tribunale di Roma a giudicare di fatti commessi in danno dello Stato, di beni e cittadini italiani, ovvero di soggetti coinvolti in quella missione,

È evidente che nessuno pensa che i pirati debbano essere trattati come storicamente avveniva in altri tempi. Il nostro Paese, che è all'avanguardia per quanto riguarda la pratica e il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, sa benissimo

certamente e assolutamente garantito. Detto questo, rimane il dato di fondo, principale e pregiudiziale a tutto il resto: questa pirateria moderna, che è un fenomeno sempre più evidente e preoccupante, va combattuta e sconfitta. Con questo auspicio il Popolo della Libertà voterà convintamente a favore di questo provvedimento.

Naturalmente il Governo, attraverso le sue strutture, sta operando sin dal primo giorno in maniera molto incisiva e con la necessaria riservatezza. Dunque, formulo insieme a lei l'auspicio che

una conferenza stampa per un aggiornamento sugli ultimi drammatici sviluppi che interessano la popolazione degli uiguri nel Nord-Ovest della Cina.

Woods, vorrei segnalare che i signori banchieri continuano la speculazione sulle materie prime.

sarà presente anche il Ministro dell'economia di questo Governo) pongano all'ordine del giorno un nuovo ordine monetario. Lo dice anche il Papa, ormai lo dicono tutti, però i banchieri continuano a speculare anche sulle materie prime. Ricordiamo che il prezzo del petrolio era arrivato a 150 dollari al barile. Le banche centrali

Nel leggerla ho trovato molti spunti per tutti gli uomini, sia fedeli che laici. Suggerirei quindi all'Amministrazione del Senato di mettere a disposizione tale testo per tutti noi.